Signor Presidente, ci troviamo qui oggi per votare l'ennesima fiducia. Eravamo preparati, onorevoli colleghi, con i nostri rilievi critici e le nostre valutazioni, a esprimere il nostro voto sulla legge di conversione del decreto legge recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca», originariamente composto di due sole disposizioni, di contenuto quanto mai lontano l'una dall'altra e ancor di più dalle ragioni di straordinaria necessità e urgenza richieste dall'articolo 77 della nostra Costituzione. Ma non è questa una novità, come non lo è il fatto che una legge di conversione assuma il ruolo di testo omnicomprensivo di disposizioni completamente slegate dal testo originario e prive prive di qualunque coerenza e organicità. Con questo provvedimento si assesta un ulteriore colpo alla credibilità delle istituzioni e del Parlamento e alla qualità delle leggi.

nella 7a Commissione se ne è fermamente convinta e da quanto tempo manca da una scuola meridionale e del resto d'Italia. Già di per sé si intendeva convertire un decreto-legge che verteva sulla prosecuzione del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (il cosiddetto programma scuole belle) sino alla data del 30 novembre 2016, mediante lo stanziamento di ulteriori 64 milioni di euro nell'anno 2016. Peccato che, dall'avvio del progetto scuole belle, invece che un aumento si sia registrata una contrazione del numero dei lavoratori coinvolti nelle attività di pulizia nonché di ripristino del decoro fisico e infrastrutturale delle istituzioni scolastiche statali. Infatti, a fronte di 19.843 lavoratori rilevati a maggio 2014, oggi ne risultano in servizio 18.148, corrispondenti a 12.846 *full time equivalent* considerando tutte le Regioni. Ciò potrebbe essere considerato un segno che questo piano straordinario, nonostante gli stanziamenti, non sta effettivamente dando i risultati dovuti? Per non parlare del parere contrario dell'Autorità nazionale anticorruzione rispetto alla proroga degli appalti dei servizi di pulizia delle scuole, che avvengono, purtroppo, senza gara. L'articolo 2 del decreto-legge, invece, prevede l'assegnazione di un contributo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute e il riconoscimento delle sue attività. Tale struttura verrà ad assumere carattere di stabilità come istituto universitario a ordinamento speciale, con profili dubbi rispetto alla copertura finanziaria, poiché la spesa quantificata nel limite di 3 milioni di euro annui è sostanzialmente destinata ad assunzioni di personale docente, tralasciando il fatto che l'istituto ha bisogno di un organico minimo che consenta alla Scuola sperimentale abruzzese il funzionamento istituzionale e l'accreditamento delle proprie attività. la relazione tecnica ben poche indicazioni fornisce in merito alle spese di funzionamento dell'istituto ed è altrettanto lacunosa in merito all'adeguatezza delle risorse previste complessivamente a copertura, cioè il 20 Oltre a questo, nell'ultima settimana sono stati presentati emendamenti dal Governo che introducono le disposizioni più disparate: dai contributi alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, all'incremento dei compensi per i commissari del concorso per docenti recentemente recentemente bandito; dall'adeguamento della normativa di accesso alle professioni regolamentate per agrotecnici, geometri, periti agrari e periti industriali all'estensione agli immigrati con permesso di soggiorno del beneficio della famosa carta elettronica con con l'importo di 500 euro per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, a eventi culturali e per l'accesso ai musei. è poi previsto il polo della ricerca nell'area dell'ex Expo di Milano. Comprendiamo l'urgenza di dare una destinazione adeguata a quel sito, ma il cosiddetto Human Technopole sembra, in tutta coscienza, sottrarre risorse ingenti alla ricerca scientifica italiana, mortificando i ricercatori e deludendo i tanti operatori scientifici onesti, coscienziosi, liberi. Pertanto, il sistema della ricerca nazionale ha bisogno non tanto di nuovi muri, di nuovi contenitori, ma di contenuti e di risorse per stabilizzare gli operatori, di investimenti in tecnologie sofisticate e di trasformare finalmente le eccellenze da episodi straordinari in ordinaria *governance* del sistema della conoscenza, delle competenze provenienti dalla nostra scuola secondaria, dalle nostre università e dai nostri politecnici. Ampia è pertanto la condivisione, per quanto ci riguarda, delle riflessioni esplicitate dalla senatrice Cattaneo e rivolgiamo l'invito al Governo a tenerne conto nell'interesse del Paese. Tutto questo viene giustificato dalla circostanza che il titolo del decreto‑legge permette di intuire che esso possa contenere disposizioni eterogenee e neanche vagamente vagamente rientranti nell'ambito della funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. Per queste ragioni e per non assecondare anche questa volta ciò che, in tutta franchezza, appare come schizofrenia legislativa, il Gruppo dei Conservatori e Riformisti negherà la fiducia al Governo. Signor Presidente, anche oggi, visto e considerato che stiamo parlando della scuola bella, della bella scuola e della buona scuola, il il Ministro non è

la scuola è una priorità di questo Governo e della maggioranza; si vede che le priorità sono altre, come è riscontrabile anche dai banchi della maggioranza praticamente vuoti. Va bene così e continua ad andar bene così. Avremmo voluto utilizzare il tempo a nostra disposizione per poter parlare di emendamenti e ordini del giorno; per poter discutere del contenuto di questo provvedimento. Avremmo voluto concluderne l'esame già ieri sera, perché alla fine, se non avessero messo la fiducia, non avremmo dovuto sprecare il nostro tempo a fare la Conferenza dei Capigruppo; non avremmo utilizzato tutto quel tempo solamente per una discussione sulla

Dico di più. Continuo a essere dell'idea che ormai la fiducia o la sfiducia ve la daranno gli italiani a ottobre e, quindi, continuate a mettere tutte le fiducie che volete. Una volta si parlava del partito della Nazione. Qui c'è il partito della cadrega, che vi darà la fiducia sempre perché è la cadrega che gli permette di darvela.

oltre che per dirvi di no per l'ennesima volta, per leggervi un documento che ci è stato mandato dagli insegnanti, in questo caso del Mida, che stanno subendo il vostro concorso. come loro vedono il vostro concorso; mi piace farvelo capire per il semplice motivo che l'anno scorso avete votato norme senza sapere di che cosa stavamo parlando. «Il concorso scuola in svolgimento fa acqua da tutte le parti. Non si pensi che sia l'ennesima lamentela dei docenti che vi partecipano. Oltre all'insensatezza di questa selezione, inutile per tutti quei docenti già valutati e abilitati, con spreco di denaro pubblico degli italiani tutti, questo concorso è la dimostrazione tangibile dell'inadeguatezza di chi, con protervia e supponenza, ha raccontato balle. Questo concorso ha evidenziato falle che, se non riguardassero la vita di migliaia di professori, sarebbero degne delle più tragicomica delle storie. Istruzioni fornite in maniera superficiale e dilettantesca sulle operazioni tecniche di svolgimento delle prove, nella formula *computer-based* di cui il ministro Giannini si è più volte fatta un vanto» «Programma Cineca costruito malamente, con criticità a livello di programmazione imbarazzanti. Centinaia di segnalazioni su errori di sistema che hanno compromesso le prove dei candidati. *Computer* che andavano in *tilt* e che non hanno consentito uno svolgimento della prova secondo uno standard minimo di sicurezza dei contenuti restituiti in fase di salvataggio dei dati. Informazioni sbagliate date da molti tecnici d'aula, totalmente impreparati e all'oscuro delle criticità insite nella piattaforma in uso per le prove. Migliaia di risposte che risultano non essere state salvate dal sistema a causa delle citate problematiche e che pregiudicheranno il risultato di altrettanti candidati. Pubblicazione di notizie contraddittorie da parte degli vari uffici scolastici regionali in merito al concorso, che hanno causato problemi ai candidati. Pari opportunità non rispettate per categorie di docenti (ad esempio mamme al termine della gravidanza o con gravidanza a rischio e docenti con gravi problemi di salute, che di fatto affrontano questo concorso senza le necessarie tutele). Distanza dalle sedi e impossibilità a svolgere il concorso vicino a casa. Notizie operative pubblicate in via ufficiale da uffici regionali che davano informazioni errate ai candidati e corrette in modo retroattivo per mettere una vergognosa foglia di fico là dove c'è materia per migliaia di ricorsi (esistono video e *screenshot* che lo dimostrano). minuti di tempo per la prova scritta per poter organizzare ben otto risposte che richiedevano ragionamento, accuratezza e un'articolazione non commisurate alla velocità richiesta. Dattilografi o professori? La progettazione didattica e la metodologia richiedono tempi più distesi. Assenza di griglie di valutazione e commissioni messe in piedi in qualche modo. In conclusione, la procedura concorsuale dimostra l'impreparazione di coloro che dovrebbero garantire trasparenza e massima efficienza, e che una volta ancora saranno sommersi da ricorsi da parte di chi, giustamente, si sente preso in giro. giro. Se questo è l'uso che il Governo fa dei soldi degli italiani, che questi ultimi sappiano e siano coscienti che la presa in giro non è solo dei professori ma anche la loro». Per questo motivo, noi non voteremo la fiducia. Vergogna!

il provvedimento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia riguarda la proroga del programma scuole belle e la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute. A proposito di quest'ultimo, va evidenziato come un intervento si renda necessario per poter garantire il protrarsi dell'attività dell'istituto che, senza i finanziamenti previsti dal decreto in discussione, vedrebbe di fatto vanificate

dovrebbero essere chiamati ad ottemperare, a maggiore ragione in un contesto come quello italiano, nel quale si è da poco provveduto a riformare un settore fondamentale dal quale dipende il futuro. Ultimamente tiene banco sempre più la questione relativa a una giusta tutela del *made in Italy*, e il nostro Gruppo ne ha fatto una battaglia anche a livello di proposte emendative, cercando di spingere il Governo a fare di più per la tutela del *made in Italy* e delle nostre ricchezze, delle potenzialità che devono trovare un giusto sbocco. Anche investire in innovazione, ricerca, alta formazione, nuove tecnologie va precisamente in questa direzione, che è una peculiarità tutta tutta italiana che ci è riconosciuta nel mondo. In un contesto mondiale in cui le distanze anche socioculturali si assottigliano sempre più, realtà come il Gran Sasso Science Institute - ma ovviamente non solo questa - vanno sostenute senza «se» e senza «ma». Le attività dell'istituto sono state inoltre analizzate dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, che ha espresso un giudizio positivo sul suo operato. Non va infine dimenticato che la nascita della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute si inserisce in un contesto dai risvolti anche economici, essendo stata immaginata all'indomani del terremoto che ha devastato l'Aquila quale uno degli strumenti per rilanciare l'area devastata dal sisma. Per quanto attiene al programma scuole belle, è chiaro che il decoro degli edifici scolastici rappresenti un aspetto determinante per la qualità e la quantità delle attività con le quali si formano i nostri ragazzi. Noi quando siamo in questa Aula del Parlamento non dobbiamo

interpretate. A seguito anche dell'accordo governativo, concluso in data 28 marzo 2014 presso il Ministero del lavoro, sono stati attivati servizi di ripristino del decoro, piccola manutenzione e giardinaggio volti alla riqualificazione degli edifici scolastici e confluiti in un progetto successivamente denominato dal Governo scuole belle della durata di venti mesi, fino al 31 marzo 2016, per un importo complessivo pari a 450 milioni, con il quale il Governo è riuscito a salvaguardare 11.000 posti di lavoro. Per quanto riguarda l'interesse pubblico, l'attivazione del progetto scuole belle ha garantito non solo la salubrità degli istituti scolastici interessati, ma anche la messa in sicurezza degli stessi, come attestato dallo stesso MIUR, che ha riportato i risultati conseguiti sul proprio sito istituzionale. Il tutto - si sottolinea - è avvenuto impegnando il 40 per cento in meno di fondi stanziati nel periodo 2010-2013

In data 8 marzo 2016 è stato firmato un accordo quadro tra Governo CGIL, CISL, Uil e il sistema delle aziende impegnate nel programma scuole belle, nel quale il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri De Vincenti conferma la disponibilità del Governo a sostenere la prosecuzione del programma scuole belle sino al 31 novembre 2016, anche mediante un apposito intervento normativo, individuando la disponibilità di 64 milioni nell'ambito del bilancio del MIUR e dando la disponibilità ad accogliere richieste di CIG in deroga da parte delle aziende per i lavoratori interessati. Il 70 per cento degli istituti necessita ancora degli interventi concordati all'interno del piano industriale contenuto nell'accordo del marzo 2014, in quanto le risorse erogate sino al momento attuale

Il progetto ha garantito il mantenimento degli standard occupazionali attraverso l'impiego dei lavoratori in nuove mansioni. Tale ultimo assunto riveste un'importanza rilevante se si considerano i gravi problemi occupazionali del Meridione, dove quelli che erano precedentemente lavoratori ex LSU e appalti storici, ad oggi da considerarsi dipendenti presso le istituzioni scolastiche, si concentrano maggiormente. Il costo, quindi, prevedibile di utilizzo alla cassa integrazione è stimabile in 45 milioni, con la decurtazione della retribuzione dei lavoratori del 20 che, sommato ai 64 milioni previsti dal bilancio del MIUR, portano a un impegno di spesa di 109 milioni. Il nostro Gruppo sta cercando di portare un contributo affinché, nei prossimi mesi, il ministro Giannini e il sottosegretario D'Onghia - qui mi sta ascoltando - evitando la cassa integrazione e trovando 21 milioni, riescano a ridare occupazione a ulteriori 11.000

ultimare questo grande progetto. Quindi il nostro è un impegno, come vi ho detto, che cerca di portare il nostro contributo per fare le leggi, le riforme le riforme affinché questo Paese si modernizzi. Sentivo dire che si cerca di mantenere la cadrega, il posto, il seggiolone. Noi, in maniera molto limpida, forse francescana, siamo qui e non chiediamo posti ma diamo un sostegno al Governo sulle leggi e sulle riforme che condividiamo. Sono altri che hanno avuto posti per dieci anni, non hanno fatto nulla ed hanno fallito!

(MpA))*. In effetti, essere ripreso da chi presenta 80 milioni di emendamenti nell'interesse della nazione, mi sembra fuori luogo, fuori tempo e fuori spazio. È da

È per questo, signor Presidente, che in maniera seria non ci appassioniamo a leggere lettere o politologi

altrettanto democratica, siamo qui rappresentanti di un popolo che costituzionalmente ci permette di lavorare per portare avanti le riforme necessarie. Lo facciamo

poco edificante il fatto che si abbiano delle opinioni *a priori* e quindi si sentano sempre gli stessi interventi, pregiudizialmente favorevoli se vengono dalla maggioranza e pregiudizialmente contrari se vengono dall'opposizione. Non è un dibattito particolarmente stimolante ed interessante. Se andiamo al merito del provvedimento, c'è una netta prevalenza degli aspetti positivi, che portano a valutare nel suo complesso il provvedimento e la questione di fiducia. Alcuni aspetti sono addirittura dovuti, anche come forma di attuazione e implementazione di quanto già approvato da questo Parlamento con la riforma sulla buona scuola. Penso all'edilizia scolastica e allo sblocco dei fondi, che vengono messi in circolo Altri aspetti - è inutile negarlo - sono problematici. Penso, in particolare, alla totale asistematicità mostrata nei confronti del sistema della ricerca, prendendo finanziamenti qua e là, finanziamenti qua e là, senza una politica chiara e identificabile in un settore così strategico. Molti hanno criticato il metodo L'apposizione della questione di fiducia effettivamente crea delle difficoltà, ma - allo stesso tempo - sposta il baricentro dal merito stretto del tema alla sopravvivenza del

e, quindi, non tale da far trapelare pericolosi intenti ostruzionistici. Noi avremmo fatto altro. Avremmo messo in campo misure urgenti per la scuola e la ricerca al fine di arginare e riparare i disastri della buona scuola,

ridurre i costi e dare certezze lavorative e salariali. Avremmo inoltre trovato risorse effettive per la manutenzione e per realizzare un piano per l'edilizia scolastica. È vero che il Governo ha già stanziato fondi, ma è chiaro a tutti che, a partire dalla poca trasparenza della mappatura, si sta cercando di investire su alcune scuole e non su altre. È urgente mettere mano alla sicurezza antisismica e antincendio (vorrei ricordare che l'obbligo delle certificazioni è stato prorogato alla bonifica dall'amianto, nonché promuovere interventi di messa in sicurezza nelle scuole a medio-lungo termine. Dal Governo sono arrivati solo annunci su risorse, ma non un piano vero che possa consentire il pieno e reale utilizzo delle risorse. Nel frattempo, l'edilizia scolastica è un'emergenza.

che si preparano a fare gli insegnanti. Avremmo presentato un piano quinquennale per l'apertura di 500 scuole dell'infanzia dai tre ai sei anni, magari con l'introduzione dell'obbligo scolastico almeno a tre anni. Come sappiamo tutti, l'istruzione dei primi anni di vita riveste un'importanza incredibile per la prevenzione contro la dispersione e gli abbandoni scolastici. Avremmo destinato risorse alle scuole dell'infanzia degli enti locali, per assumere personale e non solo quelli del sostegno, ma tutti gli insegnanti necessari a garantire diritto di accesso a tutti i bambini e le bambine nelle scuole pubbliche. Avremmo utilizzato i fondi per le scuole private per assumere insegnanti, anche quelli di sostegno per la scuola statale, in modo da garantire accesso a tutti e lasciare libertà di scelta senza oneri per lo Stato (come stabilisce la Costituzione) per chi preferisce quelle private. Avremmo presentato un piano straordinario di assunzioni per ricercatori e professori dell'università e della ricerca pubblica che sono in forte difficoltà, per togliere il blocco del *turnover*, garantendo così una migliore offerta didattica e qualità della ricerca. non avremmo istituito, forse con leggerezza, una nuova università senza le risorse aggiuntive necessarie, ma utilizzando gli stessi fondi destinati all'università e ricerca pubblica. In questi anni i tagli alla ricerca sono stati pesanti (sono stati appena tagliati 30 milioni di euro per i bandi di ricerca degli atenei) e tantissimi sono i ricercatori precari in attesa di stabilizzazione. Siete riusciti a bocciare persino gli emendamenti identici a una legge da voi firmata in attesa della migliore riforma; inoltre, come ieri è stato spiegato da più autorevoli interventi, è chiaro che la ricerca pubblica non è è una vostra priorità. Nel decreto-legge in discussione, a proposito degli appelli alla congruità di materia, è comparso uno strano articolo sull'ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità; si tratta nei fatti del recepimento della sentenza del Consiglio di Stato intervenuta per sanare scelte sbagliate. Mi chiedo però come sia stato possibile trattare un argomento così importante senza coinvolgere le Commissioni referenti e senza una discussione completa che potesse sanare del tutto le questioni ancora aperte legate alla disabilità. dimostrate di non avere alcun rispetto per il Parlamento, non solo del Senato, che impropriamente annunciate di aver chiuso, ma persino della Camera, della democrazia parlamentare, confermando già in questi passaggi il segno autoritario e oligarchico della vostra riforma costituzionale. un Parlamento che legifera solo attraverso decretazione di urgenza e fiducia, anche quando non sarebbe necessario, come in questo caso. A dire la verità, ci saremmo aspettati un intervento del Presidente del Senato a tutela del ruolo del Senato e della funzione legislativa. Il numero degli emendamenti presentati da maggioranza e opposizioni non è tale da rendere impossibile il confronto, dunque questo voto di fiducia è incomprensibile, a meno che il problema non sia tutto nella maggioranza. Qualche sospetto iniziamo ad averlo: leggendo emendamenti e ordini del giorno abbiamo la vaga sensazione

scuola, dopo meno di un anno le contraddizioni, i problemi sono tutti esplosi. Nelle scuole si respira un brutto clima, la cultura del sospetto, poca collaborazione, poco senso del lavoro collettivo. Gli insegnanti, a partire dai neo assunti (ai quali non avete concesso niente, le assunzioni sono state un obbligo imposto dall'Europa e un diritto), sono in piena competizione per il *bonus*, per compiacere il dirigente scolastico; pessima l'idea dei comitati di valutazione. Per fortuna nel Paese ci sono tante cittadine e tanti cittadini impegnati proprio in questi giorni a raccogliere le firme per i *referendum* per abrogare parti importanti della vostra «buona scuola»; una grande mobilitazione, che vede insieme genitori, insegnanti, alunni e tanti, tanti cittadini che proveranno a ricostruire una scuola statale pubblica, aperta, laica, democratica, in coerenza con i valori repubblicani e costituzionali. Confermo il voto ovviamente negativo di Sinistra

Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame affrontava nel testo originario due questioni specifiche: il completamento del programma scuole belle, per il quale si rende necessaria una proroga dei termini, e la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato di ricerca Science Institute Gran Sasso. Durante l'*iter* in Commissione sono emerse varie altre questioni del mondo della scuola rimaste in sospeso dopo l'approvazione della legge n. 107 dello scorso anno; questioni fatte emergere con la presentazione di vari emendamenti che entravano nello specifico dei problemi. La Commissione ha esaminato, poi, alcuni emendamenti del Governo, che intendevano anticipare i tempi della citata legge n. 107, per evitare che l'inizio del prossimo anno scolastico avvenisse con serie difficoltà

di considerare la scuola un settore fondamentale su cui investire per il futuro dei nostri giovani e per il futuro del nostro Paese, impegnando risorse finanziarie per affrontare le principali, annose questioni, dalla stabilizzazione dei docenti precari della graduatorie GAE e idonei al concorso 2012, al nuovo concorso, all'edilizia scolastica, all'aggiornamento e valutazione del personale, all'alternanza scuola-lavoro, per citare solo i temi più pregnanti affrontati dalla legge n. Sottolineo, poi, altre questioni che rimangono aperte, sollevate anche in alcuni interventi della giornata di ieri e discussi in Commissione, quali il distacco, limitato all'anno scolastico in corso, di docenti presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, resi necessari dalla carenza degli organici; oppure il pagamento del costo per la gestione degli edifici sede di conservatorio non più a carico delle Province, a seguito di quanto stabilito dalla legge poi ancora, il concorso per dirigenti scolastici (solo in Veneto il prossimo anno scolastico 200 istituti saranno senza dirigente e si dovrà ricorrere alla reggenza); la stabilizzazione del personale ATA. La complessità delle problematiche e la loro intersezione con altre tematiche di carattere generale costringono alla gradualità nell'adottare i provvedimenti necessari. Questo decreto-legge, sostituito dall'emendamento complessivo del Governo sui temi analizzati e votati in Commissione, si inerisce in quest'ottica. Il completamento del programma «scuole belle» non potrebbe proseguire senza una dilatazione dei tempi rispetto all'attuale scadenza, peraltro già trascorsa, del 31 marzo. Il prolungamento sino alla data del 30 novembre, con l'ulteriore stanziamento di 64 milioni di euro, consente di ampliare ed ultimare i molti interventi (oltre 17.000) ai quali è stato dato il via, con ricadute positive, oltre che sulla qualità e sicurezza degli edifici, anche sull'occupazione del personale già operante nel settore dei servizi scolastici. Intervento fondamentale è, poi, la stabilizzazione e il riconoscimento della scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute, avviato a seguito della grande calamità del terremoto d'Abruzzo per consentire una più rapida ripresa del territorio di questa Regione. Per tale Istituto, il nostro Gruppo ha presentato in Commissione un emendamento trasformato in ordine del giorno, che impegna il Governo a reperire ulteriori risorse. Valutiamo in modo positivo i temi inseriti dagli emendamenti del Governo, che affrontano altre questioni sollevate da vari Gruppi con propri emendamenti e ordini del giorno, quali le misure per l'assunzione del personale per l'anno scolastico 2016-2017, il contributo alle scuole paritarie che accolgono bambini con disabilità, le disposizioni per consentire ai docenti che svolgono servizi di supplenze brevi di essere retribuiti con tempestività e regolarità, il fondo per proseguire con i rapporti di collaborazione con il personale degli uffici amministrativi, l'incremento del compenso ai docenti impegnati nel concorso per docenti. In sede di dibattito ho posto particolare attenzione al tema delle scuole paritarie che stanno vivendo una situazione di grande difficoltà economica, che ha già portato alla chiusura di varie sezioni con l'impossibilità di garantire il servizio in alcuni Comuni, soprattutto quelli di minore dimensione. Le previsioni inserite recentemente con la legge n. 107, con la legge di stabilità 2016 e con questo provvedimento vanno nella direzione giusta, ma sono previsioni troppo modeste, non in grado di garantire la prosecuzione dell'attività di queste scuole, che pur essendo private svolgono un servizio di carattere pubblico, controllato dallo Stato con il riconoscimento della condizione di scuole paritarie. È giunto il tempo ormai di dare piena attuazione alla legge n. 62 del 2000, prendendo atto di una situazione diffusa e consolidata: queste scuole hanno cominciato a vivere l'attuale drammatica situazione con la diminuzione del personale religioso, sparito ormai ovunque. A seguito di questo, la gestione è garantita da associazioni di genitori che hanno dallo loro parte la grande risorsa del volontariato, non in grado tuttavia di garantire la sostenibilità dei bilanci.

Chiudo con una constatazione: perché anche in questa occasione, su un provvedimento che interessa la scuola, si ricorre al voto di fiducia? La 7a Commissione ha interloquito con il Governo - guai se così non fosse sia per approfondire i due temi inizialmente presenti nel decreto, sia per ampliare il campo d'azione affrontando altre questioni che affliggono il mondo della scuola. Non spetta a me difendere il lavoro della Commissione, lo faccio solo a nome del mio Gruppo, ma mi sento di dire che tutti noi abbiamo lavorato con spirito collaborativo e con disponibilità al confronto e che tranquillamente si poteva scegliere la strada del normale *iter* parlamentare anziché porre la questione di fiducia.

ci ritroviamo oggi in dichiarazione di voto sulla fiducia posta su un decreto-legge che riguarda la scuola. A luglio 2015 noi pensavamo di avere già visto il peggio, perché un Governo che porta a casa una vergognosa riforma della scuola con un colpo di fiducia non si può vedere in un Paese civile e democratico. Pensavamo di avere esaurito la nostra rabbia e il nostro dolore e invece ci ritroviamo oggi ancora con un colpo di fiducia con il quale si porta a casa un provvedimento eterogeneo per materia, e che e che ha visto l'innesto di modifiche da parte della relatrice e del Governo con emendamenti relativi a materie completamente estranee al decreto stesso.

il suo magnifico piano delle assunzioni straordinarie che ha prodotto, appunto, una situazione per la quale ci sono insegnanti che da Trapani devono prendere l'aereo per andare a lavorare a Modena, nell'organico del potenziamento, quindi a vagare come fantasmi dentro le scuole. Bene, qui si vuole porre il correttivo, si si va in deroga e si permette di chiedere l'assegnazione provvisoria. Questo in barba a tutta una categoria di insegnanti che non hanno partecipato alla fase B del magnifico piano di assunzioni straordinarie e hanno deciso di rimanere a casa loro, nella speranza poi di ottenere

Governo. Poi abbiamo gli insegnanti delle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia, quelli che la buona scuola aveva dimenticato. Eccoli che rispuntano. E non uso qui parole mie. Per parlare di questo emendamento vergognoso uso le parole della Presidente del Comitato tutela GAE infanzia, Alessandra Michielotto, che spiega come ogni ruolo che sarà tolto alle GAE,

vedrà il ricorso d'urgenza al giudice del lavoro; e sarà sollevato il principio dell'anticostituzionalità per discriminazione tra docenti che hanno parità di titoli. Quindi, siamo di fronte a un sopruso bello e buono, e il Governo ne dovrà rendere conto. Pertanto, altri conflitti, altre discriminazioni ed altri contenziosi. E questo è il Governo illuminato che abbiamo in questo Paese in questo periodo. Poi abbiamo il *bonus* di 1.000 euro a studente disabile per la scuola privata e paritaria. Trovo questa operazione vergognosa, perché si utilizza un dramma che vivono molte famiglie con le relative necessità,

nella scuola pubblica il sostegno è ancora una chimera. Nella scuola pubblica, infatti, non sono stati risolti i problemi del sostegno ai bimbi con disabilità.

tutta la disabilità va sostenuta: quella nelle scuole private e paritarie, ma anche, e soprattutto, quella nella scuola pubblica. Quindi, non si devono creare delle discriminazioni tra studenti portatori di disabilità.

con un atto di aggressione parlamentare, infila in questo decreto un emendamento che tocca una materia complessa e articolata, che non può esaurirsi in una modifica estranea

le varie sentenze del Consiglio di Stato sull'esclusione dal computo ISEE delle pensioni di invalidità, dell'indennità di accompagnamento e di ogni altra previdenza legata alla disabilità grave. Ancora una volta userò parole non mie, ma della

peggiora le condizioni per i disabili, ma crea anche una discriminazione all'interno delle famiglie che potrebbero usufruire di tutte le misure

l'apoteosi della cecità, della mancanza di visione e di strategia, della prepotenza e della presunzione, che faranno schiantare questo Governo, che colerà

Raffaele Cantone, che il 20 aprile ha detto al Parlamento e al Governo: basta con le procedure di proroga per l'affido degli appalti per la pulizia nelle scuole, perché producono dinamiche

pubblici, con il gioco delle proroghe degli appalti di pulizia nelle scuola. Noi abbiamo proposto un disegno di legge per re-internalizzare questi servizi, per ricostituire l'organico dei collaboratori ausiliari e

Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, inizierò la mia dichiarazione di voto ringraziando il presidente della 7a Commissione, senatore Marcucci,

e quella sul decreto-legge sulla scuola al Senato: due fiducie nello stesso giorno poste da un Governo che evidentemente fa fatica a tenere insieme i pezzi. Mi chiedo perché il Presidente della Commissione,

chiuso ma costruito in quel modo arruffato e pasticciato (esattamente come avviene nel mondo della scuola), ma vedremo - come ricordava qualche collega in quest'Aula - il risultato del*referendum* di ottobre.

dalle mie. Abbiamo posizioni diverse; ad esempio, noi sull'aiuto alle famiglie dei disabili e alle scuole paritarie abbiamo espresso, quando abbiamo potuto votare l'emendamento in Commissione, un voto favorevole. Naturalmente crediamo che sia giusto farlo. Allo stesso modo abbiamo presentato emendamenti di carattere diverso.

ha fatto dei richiami sugli appalti, e allora: o Cantone vale sempre o Cantone non vale mai. Naturalmente c'è superficialità, non c'è altro. È un Governo solo superficiale che non affronta i temi.

non se ne parla neanche. Siamo a questi livelli. Ma ancora, vi è un argomento che i colleghi precedentemente non hanno toccato (forse si sono dimenticati): i 500 euro. Si vota. Il *bonus* ormai va insieme alla data delle elezioni. Non mi interessa quando verranno presi i 500 euro. Si vota e allora al Governo, al *Premier* abusivo, viene una grande idea: la parola *bonus*. La associamo:

colleghi di maggioranza, cito persone, alcune a me vicine, altre lontane politicamente dal mio Gruppo: è possibile che vengano fatte delle cose che non vanno bene proprio a nessuno? Non ci si ferma a chiedersi il perché?

*(PD)*. Signor Presidente, autorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, in realtà io credo che il provvedimento che stiamo per votare sia una conferma ulteriore dell'attenzione da parte del Governo nei confronti della scuola, della ricerca, dell'educazione, della cultura in generale.

nell'ottica di considerare, appunto, l'educazione e la cultura come il vero momento di svolta e di rilancio per un sistema Paese che crede in se stesso. Lo abbiamo fatto, lo sta facendo questo Governo con fondi aggiuntivi e riforme profonde, con grande attenzione e grande sensibilità. sensibilità. Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca: questo è il tema di questo decreto-legge, decreto-legge, che è arrivato dal Governo. Non entrerò nei dettagli, visto che sono stati affrontati nel dibattito e ben spiegati, in particolare dalla relatrice. Il decreto-legge è arrivato in Commissione, in particolare con due questioni: quella cosiddetta delle scuole belle, e ci mancherebbe che non sentissimo il dovere morale e politico di proseguire quell'attività; e quella della Gran Sasso Science Institute (altrettanto importante la trasformazione universitaria di questa istituzione). Ma all'interno del dibattito si è sottovalutato un tema rilevante, forse accecati dalla vicenda e dalla richiesta del voto di fiducia da parte del Governo, credo dovuta in particolare alle alle preoccupazioni circa i tempi di conversione di questo decreto-legge. L'attività parlamentare è stata significativa su questo provvedimento. Esso è arrivato in Commissione con queste due questioni proposte dal Governo,

Il dibattito in Commissione, la presentazione degli emendamenti, le soluzioni indicate e individuate, ovviamente sempre all'interno dei temi e quindi con congruità di materia, hanno portato a un provvedimento che è molto più ricco, consistente e forte di quello che c'è stato inviato. Quindi il plauso lo faccio proprio alla 7a Commissione, ai suoi commissari, all'interlocuzione che hanno avuto in queste settimane di lavoro intenso, discutendo sulle questioni specifiche, sugli emendamenti ed esprimendosi con i voti. Certo, il Governo ha chiesto la fiducia su questo provvedimento, ma bisogna anche riconoscere che ha presentato un maxiemendamento che è esattamente la risultante della dialettica parlamentare che si è svolta all'interno della Commissione, ed ha rispettato esattamente i voti che in Commissione sono avvenuti: una cosa rilevante che credo valga la pena di sottolineare. Se era necessario provvedere ad aumentare i compensi dei commissari di concorso, la Commissione ha ritenuto di doverlo fare ed ha votato in tal secondo noi lo era - procedere verso l'assorbimento delle gare tramite la modalità interregionale, l'abbiamo fatto con un emendamento; se era importante - secondo noi lo era - dare i fondi alle scuole paritarie

se era importante affrontare la questione dell'ISEE, urgente anche in seguito a recenti sentenze, l'abbiamo fatto con grande determinazione, con voglia di confronto, ma anche con la continua ricerca tesa a risolvere questioni importanti nell'interesse del nostro Paese.

Credo che si tratti di un tema rilevante sul quale è giusto che il Parlamento si confronti; la Commissione è la sede idonea ed è a disposizione per fare questo. questo. La senatrice Cattaneo, presentando il suo ordine del giorno, ha parlato di questioni più ampie e rilevanti, che toccano l'organizzazione complessiva della ricerca nel nostro Paese. Attendo pertanto, come naturale conseguenza di tale intervento, la proposta della senatrice Cattaneo di un disegno di legge che io, insieme alle altre proposte che i commissari della 7a Commissione hanno presentato su questo tema, presto incardinerò perché credo che siano maturi i tempi per un confronto serio. Però bisogna prendere anche atto delle situazioni; bisogna prendere atto degli importanti e imponenti - li definirei così - stanziamenti anche recenti, tramite il CIPE, che questo Governo ha deciso sulla ricerca. Bisogna prendere atto della rivitalizzazione del dibattito sulla ricerca come motore di sviluppo per il nostro Paese; bisogna anche prendere atto che grazie a questo Governo finalmente l'Italia è tornata a parlare di ricerca in maniera consistente e molto concreta. molto concreta. Cari colleghi, noi del Partito Democratico continuiamo ad essere orgogliosi di votare a favore dei provvedimenti che aiutano la scuola, la cultura, la formazione, l'università e la ricerca del nostro Paese. E lo continueremo a fare. Lo facciamo oggi, esprimendo il nostro voto di fiducia lo facciamo ringraziando i parlamentari per l'attività svolta all'interno della Commissione e tutti i Gruppi per

scuole

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di

Signor Presidente, prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno, volevo proporre all'Aula l'inversione del secondo punto con il terzo provvedimento sull'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.